due giorni fa, il 12 novembre, cadeva il terzo anniversario della strage di Nasiriya, in cui trovarono la morte 19 nostri connazionali. Oggi, prima seduta pubblica del Senato successiva a quella data, credo di interpretare il pensiero di tutti voi dedicando all'inizio dei nostri lavori un momento di riflessione e di raccoglimento alle vittime militari e civili di quel tristissimo giorno che gettò nel lutto l'intera Nazione. L'Italia non dimentica i suoi figli valorosi. Le nobili parole pronunciate domenica dal Presidente della Repubblica esprimono efficacemente i sentimenti più profondi del nostro Paese verso quei coraggiosi e verso le loro famiglie così tragicamente colpite negli affetti più cari. Anche di questo siamo grati al presidente Napolitano; nelle sue parole, sono convinto, si riconosce tutto il popolo italiano. I caduti di Nasiriya, giovani vite spente mentre nella tormentata terra d'Iraq operavano con l'obiettivo di riportare pace e rinascita civile, sono luminosa testimonianza di quella fondamentale virtù civica che deve ispirare ogni cittadino, indipendentemente dal ruolo che riveste o dal compito che gli è stato affidato: il senso del proprio dovere. Il loro sacrificio ci parla anche dell'amore per la Patria e per la Costituzione e ci dice di rispettarle senza affievolimenti e senza incertezze. Facendo noi memoria di quel tragico giorno, non vogliamo solo commemorare, ma manifestare gratitudine a quegli uomini, partecipazione viva ed effettiva al dolore dei loro familiari, stima e vicinanza verso quanti si trovano, mandati dal proprio Paese, ad operare perché, in aree sfortunate e martoriate dai conflitti, i più deboli possano sperare di vivere una vita degna di questo nome e il vento della pace e della libertà torni a soffiare su quelle terre. Il Senato tornerà ad occuparsi di questi problemi in occasione dell'esame di proposte che sono state già avanzate. Il Senato della Repubblica ricorda oggi con affetto e riconoscenza i caduti di Nasiriya. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento.

di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

attraverso gli interventi dei senatori che mi hanno preceduto; cercherò pertanto di porre attenzione su alcuni aspetti che meritano ancora di essere trattati. La prima considerazione sul disegno di legge al nostro esame è stata proprio riguardo alla sua necessità e priorità.

Né in sede di Commissione, né in fase di audizione di esperti e categorie, né durante la discussione generale e l'esame degli emendamenti sono emersi convincimenti per farci credere che questo provvedimento legislativo debba essere approvato ora e subito, anche perché non mi sembra si tratti di un provvedimento rivoluzionario, e forse non ha neanche la pretesa di esserlo, proprio perché manca alcuni appuntamenti innovativi significativi. Ne cito uno per tutti: la partecipazione alle commissioni d'esame dei docenti delle scuole paritarie. Abbiamo presentato emendamenti in tal senso, tutti regolarmente respinti. È veramente difficile capire perché, dopo l'introduzione della legge sulla parità scolastica (seppure ancora molto da completare per realizzare una effettiva uguaglianza tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche private) si debba tenere in piedi questa odiosa discriminazione. Laprecisazione del ministro Fioroni in merito è servita a farci capire che dipende solo da una volontà politica: quella, appunto, di trovare la strada perché ciò possa avvenire. Ci era sembrato che in sede di Commissione si volesse aprire un dialogo sull'argomento, ma non vi è stato che un timido cenno di replica da parte della relatrice, la gentile senatrice Soliani, senza però arrivare ad alcuna conclusione positiva. Sostanzialmente, si è arrivati ad affermare che tale discriminazione andrebbe superata, ma che i tempi non sarebbero ancora maturi e che quindi deve restare. Perché? Per quale motivo, non è dato sapere. Forse perché una parte della maggioranza odia profondamente ogni espressione di libertà di educazione e quindi avversa duramente la scuola pubblica non statale? Credevo che sarebbe bastata la volontà del Parlamento per decidere in materia legislativa e che non si debba dipendere da altri, ma evidentemente per questa maggioranza non è così.

che sta lì quasi a sancire una sorta di inferiorità dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali. I primi, infatti, possono portare gli studenti all'esame di maturità, ma non possono giudicarli in quella sede. C'era da considerare anche un fatto di natura pratica. Abbiamo difficoltà a comporre le commissioni di esame e ne avremo ancora di più in futuro, quando avremo la metà più uno delle stesse composta da personale docente esterno all'istituto. Ebbene, questo rappresenta una difficoltà storicasia per la scarsa disponibilità registrata nel passato a trovare docenti disponibili, sia per i maggiori oneri economici che crescono quanto maggiore è distante il docenteche si deve reclutare per tale servizio. Con l'utilizzo dei docenti delle paritarie si potrebbero superare ambedue i problemi soprattutto nelle Regioni del Nord e nei grandi centri, dove è maggiore la presenza di docenti di scuole non statali. alle difficoltà di natura economica, mi permetto di ricordare che siamo già dovuti intervenire a valle, nel mese di luglio, a cose fatte, per coprire la spesa necessaria per pagare i componenti delle commissioni di esame di maturità. sia consentito altresì ricordare che quei fondi vennero recuperati utilizzando quelli destinati al tutorato, con il preciso impegno, espresso anche in quest'Aula, che sarebbero stati reintegrati. Sempre se non ricordo male, fu su questo presupposto e su questo impegno solenne che votammo all'unanimità la ratifica del decreto del Governo che decideva in tal senso. Non mi risulta che ciò sia stato fatto. Mi auguro di non essere aggiornato sull'argomento e che, invece, sia intenzione del Governo provvedere in questa direzione. Sarebbe altrimenti veramente deprecabile che venga smantellato un servizio altamente educativo e certamente innovativo per via secondaria e incidentale, senza un dibattito serio e una chiara presa di posizione del Parlamento. D'altra parte, mi sembra si stia procedendo in questo modo su molti altri provvedimenti connessi alla riforma Moratti. in altri termini, la riforma senza alcun dibattito politico in sede legislativa. Lo sanno i manifestanti anti- Governo, capeggiati dai «Sottosegretari del dissenso», dissenso», scesi in piazza il 4 novembre, che chiedevano la cancellazione della riforma. Lo sapevano che il Governo sta già lavorando per loro, nella direzione da loro auspicata? Forse di questo avremmo dovuto parlare in quest'Aula prima della riforma degli esami di maturità. Forse qui avreste dovuto, con chiarezza e coraggio, portare i vostri intendimenti su questa materia (la riforma in atto) e dirci sinceramente e complessivamente che cosa volevate fare, senza ricorrere a mezzucci di circostanza, con provvedimenti di natura amministrativa e, addirittura, accordi sindacali che riguardano la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Non credo di fare alcuna gratuita polemica, né inutile retorica. Credo di dire cose di buonsenso che una maggioranza organizzata intellettualmente per essere la grande svolta e il cambiamento di rotta storico dopo il quinquennio della destra oscurantista dovrebbe comprendere da sé, perché il grande governo del Paese non può essere fatto con impostazioni di tipo partigiano. Mi sembra invece che su questa materia il precedente Governo dimostrò molto più coraggio, lealtà verso gli italiani e vero interesse nel perseguire il bene comune, attuando importanti e radicali riforme del nostro apparato amministrativo di quanto siate capaci di fare e dimostrare voi. E questa mattina ne state dando una chiara conferma.

Diciamo di volere una democrazia matura, stabile, che sappia gestire le inevitabili alternanze di maggioranze diverse. In questi ultimi dodici anni si sono verificati almeno sei significativi cambi di maggioranza, due anche in corso di legislatura. Ebbene, questo non sarebbe un problema se chi governa avesse il fondamentale buonsenso di rispettare i provvedimenti attuati da chi lo ha preceduto nell'esercizio della guida del Paese. Quello che è concesso, perché doveroso, a chi subentra è di verificare, dopo un congruo periodo di tempo, il funzionamento di leggi precedentemente approvate e di apportare i necessari cambiamenti, magari con l'accordo di chi li aveva a suo tempo assunti, anche perché il popolo italiano, in quella precedente legislatura, si era espresso per avere quella legge e non altra, espressione di quella maggioranza politica di allora. E quella legge deve esserci. Ma abbiamo molte volte criticato questo vostro assurdo modo di procedere che non denota considerazione per gli amministrati e i cittadini italiani in genere. Nella discussione del provvedimento in esame avevo sottolineato come questo vada ad aumentare quel clima di generale incertezza che purtroppo regna nella scuola italiana, sia fra i docenti, i presidi, o dirigenti scolastici che dir si voglia, sia fra gli studenti, sia fra le famiglie. Quello che viviamo sembra essere, per suo carattere costitutivo, il tempo delle incertezze, ma ritengo che questo non giovi a nessuno: incertezza sulla famiglia e sulla sua stessa natura, come i recenti accadimenti verificatisi alla Camera dei deputati sulle unioni di fatto stanno a dimostrare; incertezza sulla scuola, i suoi percorsi formativi e sul futuro lavorativo che da questi percorsi dovrebbe derivare. Non mi sembra che debbano essere appunto questi i caratteri costitutivi della crescita dei nostri ragazzi. Non meritano un Paese che non sa dare certezze. Al di là di tante inutili formulazioni di natura pedagogica e di strampalate teorie, che hanno infelicemente dominato in questi ultimi anni, credo che i nostri ragazzi oggi, come noi qualche decina di anni fa, abbiano bisogno soprattutto di certezze. Ebbene, questa ulteriore riforma va un po' ad aggravare questo stato di confusione e incertezza che purtroppo domina nella scuola italiana da troppi anni. Negare ciò, e non prenderne atto, è pura miopia politica e culturale.

quella del controllo e della verifica sull'attività dell'Esecutivo. Invece in Commissione non ho avuto alcuna risposta in merito. Era evidente che, sotto un'apparente intenzione di dialogo, la volontà vera è quella di approvare rapidamente questa legge e, magari, anche di portarla in immediata applicazione (di quest'ultimo aspetto parleremo fra poco). È chiaro, invece, che si vuole continuare a legiferare, magari anche con grande frequenza, nella stessa materia e direzione, perché si è convinti che la società muti tanto rapidamente da dover toccare e ritoccare in continuazione, attraverso la legge, le regole della vita civile e amministrativa degli italiani. Questa ossessione ideologica, in base alla quale tutto deve essere disciplinato, ogni spazio di libertà gentilmente concesso dallo Stato deve poi essere regolamentato fino all'asfissia, è un modo vecchio di vedere la società *(Applausi dai Gruppi* delle energie culturali ed educative del nostro Paese, che sono ancora, grazie a Dio (non uso un'espressione fatta), molte e vitali. Siamo il Paese con il maggior numero di leggi in Europa e forse nel mondo, ma non per questo funzioniamo meglio di altri; anzi. Nella scuola, in modo particolare, dovremmo avere una prudenza - direi - eccessiva, prima di intervenire in alcun modo. Dovremmo lasciare che la scuola lavori in serenità e in continuità nella certezza del domani e che non subisca improvvisi e continui cambiamenti. Dovremmo aspettare, magari, un intero ciclo didattico, visto che tutti i livelli e i periodi scolastici hanno subito profonde e radicali riforme, dalle materne alle superiori, fino alla stessa università. Dovremmo riguardare tutta questa legislazione e verificare, senza cecità ideologiche e liberi da qualsivoglia questione di tipo corporativo o sindacale (di per sé legittima), la coerenza normativa e l'effettiva funzionalità di tutte le riforme messe in campo fino ad ora; vedere, ad esempio, se ogni percorso aggancia bene il successivo, se c'è un'adeguata continuità, se ci sono inutili ripetizioni. Forse, fatto tutto questo, riusciremmo a capire quale possa essere la migliore prova finale di questo processo formativo: l'esame di maturità. Potremmo anche arrivare alla conclusione che esso non serva a nulla, autorevole opinione che sta sempre più prendendo campo, o che debba essere ancora più rigoroso e selettivo dell'attuale; ma lo diremmo dopo una seria e puntuale verifica. Ritengo doveroso, per tutto questo, chiedere una riflessione più attenta ed approfondita. La stessa motivazione fondamentale per cui la legge viene presentata è quella di garantire maggiore rigore e serietà per questo tipo di esame e ridargli più dignità e significato. Il fenomeno Il fenomeno che viene indicato come negativo è l'eccesso dei diplomati, soprattutto nelle scuole paritarie, dove risulterebbe più agevole il meccanismo dei cosiddetti «ottisti», cioè l'accesso diretto dal quarto anno all'esame di maturità in presenza di uno scrutinio che assegna almeno otto decimi su ogni materia.La relatrice Soliani denuncia opportunamente come questo fenomeno abbia portato, in alcune scuole, alla promozione di quasi intere classi del quarto anno alla maturità. Per rispondere a ciò, il disegno di legge prevede un aggravamento di condizioni per l'accesso a questa abbreviazione del percorso didattico. Avevamo seguito questa linea, inserendo l'obbligo di non aver mai conseguito debiti. Sempre sulla linea di un maggior rigore, avevamo proposto, insieme al collega Buttiglione, che l'esame orale, il colloquio, potesse spaziare su tutto l'arco del percorso formativo e non solo sull'ultimo anno, magari mantenendo un giudizio e una valutazione prevalente sulle materie dell'ultimo anno. Ma ambedue queste proposte non sono state accolte, se pur apprezzate. Resta comunque il fatto che l'esame di maturità è la conferma di un percorso di cinque anni fatto ad un giovane che si conosce, non è la prova di concorso di un candidato fra mille che si vede per la prima volta. Mi permetto di ricordare che la scuola vincente è quella che riesce a portare uno studente alla fine del percorso didattico; così vorremmo che fosse anche per l'università, che invece perde troppi iscritti negli anni successivi al primo. Già è molto, troppo alto il numero dei respinti negli anni precedenti al quinto. Già è fin troppo maturata una sorta di mentalità produttivistica in parte del corpo docente, che lo porta ad esprimersi in termini sindacal-aziendali: «il ragazzo mi lavora, mi produce o non mi produce». Non credo vada alimentata questa tendenza culturale accrescendo la facilità alla bocciatura, soprattutto nell'ultimo anno di corso; questa eventualità dovrebbe essere estrema e marginale, come attualmente è. Credo che anche un operaio chiamato a rispondere della sua capacità produttiva e lavorativa debba essere valutato nel complesso della sua personalità e non solo con i numeri e la quantità, visto che è un essere umano e non una macchina; a maggior ragione un giovane studente dovrebbe essere valutato sul complesso della sua maturazione, delle sue capacità e della sua formazione culturale. Per tutto ciò, forse potevate limitare l'intervento legislativo su poche questioni, senza dare enfasi eccessiva a questa riforma, voluta, sembra, con grande determinazione. Mi auguro che maturi nella maggioranza una volontà concreta di dialogo e una più profonda disponibilità ad un confronto che produca qualcosa di più di ciò che è accaduto in Commissione. Mi è sembrato infatti che, al di là di tante buone considerazioni di principio sulla necessità di un dialogo franco e produttivo fra maggioranza e opposizione, non ci sia stata una grande disponibilità al compromesso e solo pochissimi emendamenti siano stati accolti, rarissimi quelli accolti nella loro integralità. Se i nostri appelli ad un serio ripensamento sulla necessità di questo provvedimento cadranno nel vuoto - come prevedo - si pone immediatamente un'altra questione: quella dell'applicazione della legge. Sui tempi di applicazione il collega Davico aveva proposto un opportuno emendamento che è stato regolarmente respinto. Personalmente ho posto, solo in corso di discussione, la questione dell'inopportunità dell'applicazione ad anno scolastico avviato. Non ho ricevuto nessuna risposta esplicita che motivasse la necessità di applicare da subito la legge. Vorrei su questa problematica dare voce a un genitore che mi ha cortesemente scritto, e che in verità non è stato l'unico; credo che possa rappresentare bene il sentimento - e non solo quello, anche il convincimento - della quasi totalità dei genitori e degli studenti su questo argomento: «Mi sembra indiscutibile la profonda ingiustizia e l'evidente errore giuridico che verrebbero commessi ove si ritenesse di applicare la riforma dell'esame sin dall'anno scolastico in corso; è davvero contrario a giustizia pensare di poter cambiare le regole del gioco quando il gioco è già iniziato; l'intenzione manifestata dal Governo in tal senso sta creando oltretutto uno stato di assoluta incertezza e nei docenti e negli studenti; la modifica ad anno iniziato troverebbe tutti impreparati e darebbe luogo ad incredibili improvvisazioni; ciò appare assai ingiusto rispetto all'affidamento che studenti e famiglie hanno fatto sulle caratteristiche della legislazione vigente al momento in cui hanno iscritto i figli all'ultimo anno scolastico. E' decisivo in proposito anche ricordare che l'esame non è un concorso a se stante, ma è conclusivo e fa parte, come un tutt'uno, dell'ultimo anno scolastico, che è già iniziato e le cui regole non possono essere spezzate. Senza contare che i privatisti si troveranno di fronte ad un complesso di regole abbastanza innovativo rispetto alla vigente normativa: anche per loro vale lo stesso discorso di giustizia sostanziale: non si possono cambiare le regole ad anno iniziato in un tempo molto prossimo all'esame, quando è presumibile ritenere che il candidato si sia già messo a studiare». Il carattere di buonsenso di queste parole è evidente

Un'altra questione che avevo sollevato era quella dello scrutinio di ammissione all'esame. Avevo proposto che l'ammissione fosse possibile anche in presenza di un massimo di tre materie con valutazione negativa. E' evidente che essendo questo consentito per tutto il percorso didattico nel passaggio da un anno di corso all'altro, non si capisce perché non debba essere possibile anche in sede di ammissione all'esame di maturità. Non è sufficiente delegare il Governo in questa materia, come il disegno di legge prevede. Di fronte a queste, credo significative, motivazioni ci aspettiamo una qualche risposta positiva da parte della maggioranza e del Governo sulla base della quale faremo dipendere la nostra decisone di voto.

e delega il Governo a intervenire per costruire regole e esperienze su una materia inedita nella pratica della scuola italiana, cioè il raccordo tra scuola e università. Una visione complessa dell'orientamento, che mira a superare la separatezza tra scuola e università di cui fanno le spese in genere gli studenti, anche i migliori. Il tempo dedicato a questo provvedimento in Aula è stato scarso, frammentato e spezzettato. Ciò non ha certamente incentivato l'attenzione delle senatrici e dei senatori. Eppure, questo provvedimento è importante e atteso dal corpo vivo della scuola. La mancanza di attenzione politica e di tensione testimonia il fatto che molti giornalisti e opinionisti politici parlano della scuola come argomento di cui sono in qualche modo informati. Essi, però, non hanno mai la curiosità e la passione per mettere a fuoco i problemi veri di questa in relazione all'oggettiva centralità strutturale che il sistema d'istruzione assume nella vita di un Paese, in quella di uomini e donne, soprattutto oggi in quella che tutti definiscono la società della conoscenza. Quattro anni fa uno sciopero generale della CGIL-Scuola criticava la legge finanziaria che modificava la composizione delle commissioni degli esami di maturità rendendole tutte interne agli istituti scolastici. Il pretesto fu il risparmio economico ma il risultato immediato fu una dequalificazione di quell'esame, un colpo di spugna all'idea del suo rigore e del suo valore. Si è avviato un processo che ha inficiato la rilevanza sociale di quel momento e del suo senso nella biografia individuale dei giovani, decostruendo un passaggio codificato nell'immaginario collettivo come prova che offre ai giovani l'occasione di misurarsi con il mondo degli adulti a partire dalla sintesi della loro vita scolastica. Il risparmio era una giustificazione di facciata; in realtà, esiste un nesso fra riduzione a rito vuoto e privo di senso dell'esame di maturità e l'obiettivo a lungo termine della abolizione del valore legale del titolo di studio. obiettivo è iscritto nelle filosofie delle politiche scolastiche neoliberiste, espresse in Europa da Maastricht in poi, ma elaborate assai prima dalla tavola rotonda degli industriali europei. hanno parlato di decostruzione e definanziamento della scuola pubblica, di aziendalizzazione del suo funzionamento, di riduzione dei docenti a semplici specialisti delle tecniche didattiche, divisi fra loro da rapporti gerarchici e di subalternità. insomma, di dequalificazione della scuola pubblica. Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia ed ex vice presidente della Banca Mondiale, ha chiarito, a partire dalla sua vasta esperienza, che il neoliberismo non è interessato a sostenere i sistemi di istruzione pubblici e di qualità. Tanto è vero che la stessa Banca Mondiale pone come condizione per la concessione di prestiti ai Paesi del Sud del mondo che le somme stanziate non vengano utilizzate per l'alfabetizzazione e l'istruzione.

dell'idea del sapere come diritto universale. Oggi non solo sosteniamo che il sapere è un diritto universale, ma lo affermiamo con parole più appropriate e adeguate all'analisi politica del tempo. Il sapere è un bene comune.

punto di forza di questo testo di legge è il maggiore rigore con cui si articola l'impianto dell'esame, non solo perché la commissione è composta da una maggioranza di docenti esterni, il che assicura il carattere di terzietà e neutralità, che una commissione di esame di Stato deve avere, ma soprattutto perché si ripristina il giudizio di ammissione e la necessità per gli studenti di saldare i debiti formativi degli anni precedenti. Questo non viene preteso all'interno di una visione nozionistica dei saperi e punitiva dei giovani, ma si manda loro un messaggio di fiducia e di valorizzazione delle loro capacità e del loro impegno. Infatti, in tutte le attività umane quando le aspettative sono alte, i risultati salgono; quando invece gli obiettivi si abbassano, tutto si appiattisce nell'indifferenziato e nella deresponsabilizzazione. Insomma, puntiamo alla qualità. Per questo attribuisco una grande importanza alla definizione di esame che viene articolata nel testo. testo. Ritengo tale definizione un segno positivo di discontinuità con l'idea che di questo esame ci si era fatti nel passato grazie alla riforma Berlinguer e alla riforma Moratti Si ritorna a nominare la cultura, la capacità critica, cioè un sapere alto e generale che comprende certamente come elemento costitutivo l'informazione, la nozione, l'abilità, la competenza, l'uso dei linguaggi, ma li supera, coinvolgendo la soggettività, la persona nella sua interezza e il suo rapporto non subalterno con la storia e con il mondo. Un sapere, insomma, che ha a che fare con la libertà e con la responsabilità. Ci sono punti in questa legge che non condividiamo, in quanto li riteniamo arretrati e non opportuni; abbiamo tentato di emendarli con un lavoro aperto e leale in Commissione. vi è la riesumazione dell'INVALSI per disporre modelli per la terza prova e per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in uscita dalle quinte superiori. Questo è in palese contraddizione con l'autonomia didattica delle scuole che fonda la logica della terza prova; è un invito esplicito all'esercizio della pigrizia e della genericità, vista la complessità, la fatica e l'aderenza al piano dell'offerta formativa che l'elaborazione di questa prova comporta. Ma soprattutto si tratta di una immeritata rimessa in gioco dell'INVALSI: se è vero, come noi sosteniamo con forza, che è assolutamente necessaria una valutazione di sistema, essa non può essere proposta senza una soluzione netta di continuità dell'azione dell'INVALSI

impianto culturale, metodologia scientifica, rapporto non autoritario e di comando con le scuole. Pensiamo poi che sia scorretto pedagogicamente e perdente in prospettiva aumentare il peso dei crediti formativi del *curriculum* scolastico nel punteggio finale dell'esame; anzi, pensiamo che in prospettiva dovrebbero addirittura diminuire, rivalutando il valore del giudizio di ammissione e dell'esame in sé. in sé. La storia scolastica pregressa, infatti, non può diventare per lo studente una gabbia da cui è difficile emanciparsi. Non si coglie che il dato tipico della vita degli adolescenti e dei giovani è la discontinuità e il mutamento; in tal si premiano solo le carriere scolastiche regolari e diligenti e non tipi diversi di intelligenze e di capacità, senza tener conto che il successo scolastico regolare è ancora inevitabilmente legato al censo ed al contesto di provenienza. Per finire, pensiamo che dare ai candidati esterni la possibilità di sostenere gli esami di maturità nelle scuole private paritarie sia una forzatura indebita della legge di parità, attribuisce a quelle scuole una funzione di accertamento e certificazione che compete allo Stato e quindi alle scuole statali. Una convinzione che nulla ha a che fare con il cosiddetto statalismo, ma con la necessaria e logica distinzione fra natura e carattere pubblico e funzione. Se cade questa distinzione, le scuole paritarie diventerebbero articolazioni dello Stato. Stato. Surrettiziamente, dunque, a partire da un elemento marginale dell'esame di maturità, si opererebbe una modifica di tale portata. Mi auguro comunque che questo testo, nel complesso positivo,

n. 960 piomba in un momento particolarmente delicato in Italia, un momento in cui la finanziaria, e non soltanto essa,

in un momento nel quale, come il nostro Capogruppo in Commissione di merito, senatore Valditara, ha già dichiarato, la scuola sta soffrendo una crisi eccezionalmente ampia,

che, per risparmiare risorse, prevede che i docenti dovranno bocciare di meno; come se presupponessimo che i docenti possano essere in grado di stabilire *ab* *ovo,* senza

e ci porterebbe anche, lo dirò nel corso dell'intervento, a uno scadimento di quei titoli di studio sui quali stiamo operando. Il disegno di legge mira a intervenire sugli aspetti rimasti problematici. Nell'articolazione del sistema di verifica dei titoli di studio e lo stesso pretende, come si legge nel testo della relazione (alla quale, devo dare atto, ha lavorato con grande solerzia la senatrice Soliani, aperta al dibattito e al confronto in ogni occasione con il nostro e anche con gli altri Gruppi), di garantire credibilità e dignità all'esame di Stato, non considerando che tali termini non possono derivare agli esami di Stato da parametri parziali ma da un complesso di giudizi. È come se mettessimo in dubbio dal 2001 fino a oggi - il 2001 è l'ultimo anno della composizione mista della Commissioni - la credibilità e dignità di coloro i quali quell'esame hanno superato.

Ma veniamo alla formulazione definitiva, così come arrivata in Aula, del disegno di legge n. 960. La senatrice Soliani riporta nel testo della sua relazione alcune parole,

È un parere nobile quello di Benedetto Croce, ma vorrei anche ricordare che insieme a Benedetto Croce proprio in quegli anni un altro senatore e un altro filosofo

quei momenti tragici che Pansa ha illustrato benissimo nei suoi ultimi scritti. Di Giovanni Gentile si è invece ricordato il ministro dell'istruzione Fioroni nella sua relazione al disegno di legge che oggi discutiamo, riconoscendo in quello della riforma gentiliana il modello organico di esame di maturità, coerente con le tradizioni della cultura italiana. Sono parole tratte dalla sua relazione che spero non gli siano di nocumento, così come non furono di nocumento a Giovanni Gentile. Gentile. Giovanni Gentile aveva pubblicato nel 1912, prima della dichiarazione di Benedetto Croce, un testo di capitale importanza a cui si ispira la riforma globale attuata nel 1923 dallo stesso Gentile,

le frasi di Croce, ma mi permetto, anche seguendo le indicazioni del ministro Fioroni, di ricordare quanto Giovanni Gentile disse sulla riforma della scuola e sull' esame di maturità, appena citato. Ricordo anche che quella riforma della scuola, attuata mediante legge delega al Governo in soli diciotto mesi, dall'ottobre 1922 al luglio 192,4 durante i quali il filosofo amava essere più filosofo che senatore del Regno - ricoprì la carica di Ministro della pubblica istruzione, fu una riforma complessiva, a cui in questa stessa Aula, da questi stessi banchi

«Io non avrei potuto propormi di toccare soltanto la scuola elementare o di riformare solamente una parte dell'istruzione media nel 1923, rinviando al 1924 il resto. Il programma doveva essere compiuto entro il 31 dicembre 1923». egli mise in conto che una riforma soltanto di un passaggio poteva apparire parziale e non essere consequenziale ad un disegno più ampio. Anzi, potuto avvenire, riformando soltanto un passaggio nel *cursus* scolastico, di trovare quei momenti in discrasia con altri momenti del *cursus* degli studenti e anche dei docenti. Quell'esame di Stato poteva assicurarsi credibilità e dignità perché segnava la fase conclusiva di un processo e di un itinerario che, non diversificandosi da un itinerario speculativo dello spirito umano e, sulla base di un sistema filosofico e pedagogico di vastissima la scuola è: «non diminuzione e prostrazione dello spirito, non meccanizzazione artificiale delle categorie della vita, ma la più chiara celebrazione di quello..., e che perciò vi si deve parlare quello stesso linguaggio che l'uomo parla in famiglia e nella società, o nei libri, ove concentra e potenzia le forze interiori dell'animo suo;» una scuola, aggiunge ancora Gentile, dove «si deve respirare la stessa aria del mondo al di là dalle pareti della classe», come poc'anzi si ricordava dai banchi dell'opposizione, «quell'aria frizzante e vivificante che è la gioia e la serietà della vita nel suo spontaneo rigoglio. e questo è il punto che riguarda veramente il problema che ogni legge che ad essa si riferisca deve tenere in considerazione - «che deve contentarsi di stimolare, additare una luce lontana, una meta alta, non pretendere pappagallesche ripetizioni e virtuosità disquisitorie di dottori in erba. La via del sapere sincero è lunga; ed è molto se nell'adolescenza, quando i nostri maestri hanno cure speciali pel nostro spirito, noi c'invogliamo di

Dobbiamo perciò capire e interrogarci se le scuole parificate - a proposito dell'intervento di chi, dalla maggioranza, mi ha preceduto - siano non da sopprimere o privare della partecipazione di pari rango alle funzioni della scuola statale, quanto invece da bonificare nelle gestioni - questo sì - e nei controlli, perché talvolta abbiamo illeciti e abusivismo negli interessi privati che, in diversi casi, queste conservano. Non vi è dubbio che anche nel mondo della scuola privata vi sia un pianeta di giustizia, di cultura e di legittimità che non possiamo assolutamente censurare. Dobbiamo chiederci e sapere anche se le scuole statali non necessitino di maggiori e più intensi controlli in tutti i settori (i fatti recenti lo confermano, anche se sfociano nel *glamour* e nel pettegolezzo, come lei, signor Presidente, avrà letto questa mattina), da quello della gestione degli uffici e del personale amministrativo a quello dell'intero corpo docente, verificarne la funzionalità, le garanzie e anche la trasparenza con cui operano nei settori di competenza. La scuola di Stato, che la maggioranza ritiene *tout* *court* senza macchia e senza dolo, è anche quella che produce la fuga degli studenti verso gli istituti privati. Secondo voi, per un vezzo delle famiglie o per un senso aristocratico della vita

sembra ancora che lo spettro, non dico il fantasma, ma la memoria illuminata di un Ministro storico che, in diciotto mesi, riformò non solo l'esame, ma l'intero ordinamento, dalla scuola all'università, ci possa fornire uno spunto di riflessione che intendo proporre a quest'Assemblea, che non deve dividerci secondo il ruolo di maggioranza e di opposizione. In questo disegno collega Soliani, tutti abbiamo svolto un ruolo propositivo e - ripeto - le do atto della sua assoluta coerenza e della correttezza con la quale ha condotto i lavori. La riflessione è la mi farebbe piacere se anche lei la ascoltasse per una vanità non mia, ma di Giovanni Gentile: «Tutta la scuola è vita dello spirito che lega uomo a uomo, coi viventi, coi morti e coi nascituri, e non lega solo l'uomo all'uomo, ma l'uomo al mondo, che è tutto l'essere stesso dell'uomo». *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sistema scolastico nazionale è da sempre al centro del dibattito politico tra le classi dirigenti e occupa un posto di rilievo all'interno dell'organizzazione dello Stato. Le ultime legislature confermano questa attenzione riformatrice nei confronti del settore della scuola. Nella XIII legislatura abbiamo avuto la legge Berlinguer, nella XIV legislatura la riforma Moratti e in questa XV legislatura, benché appena agli inizi, non poteva perciò mancare un provvedimento che mettesse nuovamente mano alla scuola. Il provvedimento che ci troviamo qui a discutere, però, a differenza di quelli del recente passato si limita semplicemente a modificare un singolo aspetto del sistema scolastico: l'esame di maturità. Si ha, pertanto, l'impressione di assistere ad un anomalo ciclo di corsi e ricorsi che vede prima il Governo Berlusconi eliminare la commissione esaminatrice mista, prevedendo al suo posto una commissione esaminatrice interna, e poi il Governo Prodi ripristinare la vecchia commissione mista, sia pure con il sottinteso di smantellare al più presto l'intera riforma Moratti, magari attraverso la finanziaria. Il rischio è di giocare tutto sul campo della politica, degli interessi di parte, perdendo di vista ciò che è davvero importante, ossia congegnare un buon sistema scolastico, al di là delle contese politiche. Questo è un punto sul quale soffermarci, perché solo un buon sistema scolastico può effettivamente formare una buona classe dirigente. Un limite sostanziale del disegno di legge delega in esame è rappresentato dal fatto che il Governo tratta il settore dell'istruzione come un terreno di scontro ideologico tra schieramenti politici, senza considerare che la scuola rappresenta invece un patrimonio comune e senza considerare che le problematiche ad essa inerenti debbono essere risolte con l'apporto e la condivisione di tutti coloro che hanno responsabilità politiche. Purtroppo, il Governo Prodi è unicamente intento a smontare le riforme approvate dalla precedente maggioranza, preda - com'è - di una cupa ossessione maniacale che lo porta a cancellare qualsiasi traccia del riformismo del centro‑destra, preda - com'è - di un sogno controriformista che danneggia il Paese e soprattutto i giovani di questo Paese. La *ratio* che muove il Governo Prodi è d'altronde quella di un antiberlusconismo *a priori*, di un antiberlusconismo ideologico, al quale sacrificare tutto, persino la ricerca di soluzioni legislative nuove, persino le residue velleità riformatrici di un Esecutivo consegnatosi totalmente alla sinistra massimalista. L'altro limite sostanziale del disegno di legge delega in esame consiste nel fatto che è difficile pensare pensare e realizzare seriamente una riforma dell'esame di Stato al di fuori di un più generale disegno di riforma della scuola, al di fuori di una valutazione sui percorsi universitari le cui modalità incidono - non potrebbe essere altrimenti - sulla natura e il senso stesso dell'esame di maturità. Come non vedere, ad esempio, che la laurea di tre anni e la conseguente struttura di laurea del tre più due ha diminuito il senso e l'importanza dell'esame di maturità? Affrontare un disegno di legge come questo è quindi come intervenire sulla singola parte di un insieme, senza avere a riferimento un'idea di cambiamento dell'intero sistema; è come preferire ad una riforma una mezza riforma. A dimostrazione della scarsa importanza o, meglio, della mezza importanza, che nei atti il Governo Prodi assegna alla scuola, vorrei ricordare che nel suo programma il Governo Prodi propugnava investimenti straordinari e risorse aggiuntive per il sistema scolastico e che però, proprio su questo punto, esso è oggi già sconfessato dall'attuale manovra finanziaria, la quale - com'è noto - contiene invece tagli al settore della scuola e, in particolare, al settore dell'università. Passando ora ad illustrare più da vicino il provvedimento all'esame dell'Assemblea, ovvero l'Atto Senato n. 960, recante la riforma degli esami di maturità, vorrei sottolineare, in quanto membro della Commissione istruzione, il lavoro svolto in quella sede nell'intento di migliorare il provvedimento, perlomeno laddove era possibile. I punti salienti e centrali del disegno di legge governativo riguardano - come abbiamo detto - la reintroduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato e la composizione interna delle commissioni d'esame. La composizione mista delle commissioni non è peraltro una novità: fu introdotta nel 1997. Tali commissioni erano composte in modo da assicurare un'equa suddivisione tra membri interni e docenti esterni, comprendendo tra questi ultimi il presidente. La successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ovvero la legge finanziaria del 2002), è intervenuta sulla formazione di tali commissioni giudicatrici, disponendo la presenza di soli membri interni e di un presidente esterno che fosse comune a tutte le commissioni dell'istituto scolastico. Tali modifiche erano giustificate dal contenimento della spesa pubblica e atte ad assicurare un certo grado di autonomia ai docenti delle singole classi nella valutazione finale dei propri allievi. Si dice però che un ritorno alla commissione esaminatrice mista serve a recuperare serietà. Ma come conciliare questo parziale e limitato recupero di serietà con i provvedimenti messi in atto dal Governo, attraverso la finanziaria, per aumentare del 10 per cento il numero degli studenti promossi, in modo da avere meno ripetenti, meno classi e meno costi? Cos'è? Una serietà al risparmio? Oppure una serietà ad intermittenza? Del resto, cosa potevamo aspettarci da un Governo il cui Presidente del Consiglio proponeva, in campagna elettorale, di riportare addirittura la serietà al potere? L'abbiamo vista questa serietà! È la serietà di un Governo che marcia in piazza contro se stesso o contro parte di se stesso e che, su qualsiasi argomento, è sempre e comunque contro parte di se stesso. Probabilmente, quella prodiana, è una mezza serietà al servizio di un mezzo Governo. L'attuale disegno di legge governativo si pone, inoltre, l'obiettivo di individuare elementi di raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale, rafforzando soprattutto l'orientamento e prevedendo comunque incentivi economici a favore della scelta di alcune discipline. Si tratta di obiettivi condivisibili, certamente, ma che erano già alla base della riforma Moratti. In effetti, a ben guardare, le proposte del Governo Prodi in materia di istruzione non si discostano molto dall'apposita normativa vigente, tanto da rappresentare - scusate la franchezza - una mezza innovazione. Vorrei infine sottolineare il mio apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione dai senatori dell'opposizione. Un lavoro serio, improntato a un dibattito costruttivo sul merito del provvedimento e caratterizzato da un clima di leale confronto, di cui devo rendere merito alla presidente della Commissione, la senatrice Vittoria Franco. Tuttavia, il testo che approda oggi in Aula presenta ancora forti criticità e contraddizioni che, a mio avviso, non possono e non debbono essere sottovalutate. Mi riferisco, in particolare, alla presa di posizione del Governo circa le scuole paritarie, degradate a scuole di serie B. Infatti, il provvedimento governativo prevede uno sbarramento per i privatisti che - trattati alla stregua di figli di una scuola minore potranno sostenere l'esame solo presso le scuole statali e non più presso le scuole paritarie. Un fatto inaccettabile e in palese contrasto sia col dettato costituzionale sia con la legge n. 62 del 2000 che pongono invece sullo stesso piano le scuole statali e paritarie. A ben vedere - e concludo - il disegno di legge in esame riassume in sé il carattere del Governo Prodi: un Governo la cui impronta è tutta ideologica e che, non potendo realizzare riforme, a causa di contrasti interni, si accontenta delle mezze riforme, delle mezze misure, della mezza innovazione e della mezza serietà. Un mezzo Governo, insomma, che l'opinione pubblica, anche se non costituita in commissione esaminatrice, ha già bocciato.

riformare per la terza volta in tre legislature gli esami di Stato, come ci accingiamo a fare, può apparire come un accanimento contro la stabilità del sistema scolastico; non è così e il mondo della scuola l'ha capito. Questa riforma è necessaria: è necessaria per gli elementi di maggior rigore e serietà che introduce, è necessaria per il collegamento istituzionale più stretto che viene previsto attraverso azioni di orientamento agli studi di alta formazione, utili anche per ridurre la dispersione universitaria.

Ha fatto bene la relatrice, senatrice Soliani, ad insistere su questo aspetto, facendo riferimento più volte alla parola «futuro»: il futuro dei giovani, dell'Italia dell'Europa. Non è retorica, è preoccupata fotografia della realtà che ci dice che stiamo correndo il grave rischio di restare indietro, troppo indietro, rispetto alla domanda di istruzione e di formazione che la società della conoscenza richiede. Noi sappiamo, e ne siamo orgogliosi, che il nostro sistema di istruzione dispone di punte di eccellenza, di grande eccellenza, ma è anche vero che esistono aree vaste di inefficacia, come rivelano i dati delle agenzie di valutazione internazionale, come l'OCSE, che ha parlato di un grado di istruzione degli italiani decisamente più basso della media europea e di una difficoltà di comprensione in matematica e lettura da parte di una percentuale elevata dei nostri quindicenni: non possiamo restare indifferenti rispetto a questi dati e a queste statistiche. La 7a Commissione, lo voglio annunciare anche qui in Aula, ed aspettiamo l'autorizzazione del Presidente, ha varato all'unanimità un'indagine conoscitiva a partire dai dati OCSE per capire per meglio aiutare la scuola e le istituzioni pubbliche a trovare i rimedi più efficaci. La riforma degli esami di maturità, oggi all'esame di questa Assemblea, è uno, solo uno, dei molti tasselli da costruire. Capisco le obiezioni sollevate dai colleghi: dobbiamo riformare la scuola superiore e abbiamo ancora molto da fare, riempiendo di contenuti i due anni in più di obbligo scolastico, riconoscendo più potere alle autonomie scolastiche. molto da fare per consolidare la missione di maggiore efficacia del sistema scolastico e, tuttavia, porre oggi all'attenzione del Parlamento la riforma degli esami di Stato ha un grande rilievo, ha un'importante ragion d'essere; questa riforma presente, credo, e spero, che il fatto che negli anni si sia attenuato il valore di un rito di passaggio che produce un salto di maturazione e di acquisizione di responsabilità nei giovani ha significato un abbassamento generale del livello di istruzione e della qualità dell'apprendimento. Occorre ritornare a dare ad esso il valore pedagogico ed anche simbolico che aveva in origine. Il maggior rigore previsto dal disegno di legge in esame, rispetto alla normativa attuale, va in questo senso e non c'è dubbio che sono previste norme più rigorose: la commissione d'esame composta per metà di commissari esterni;

per addestrarli a vivere e a lavorare in una società nella quale prevarrà, e dovrà necessariamente prevalere, sempre di più, il merito. Nella società della conoscenza non può che essere il merito a essere premiato. Non si tratta dunque di un rigore fine a sé stesso, vorrei rassicurare i giovani studenti e le loro famiglie: è per il loro bene, per prepararli meglio al loro futuro in una società che muta e che avrà, sempre di più, il suo perno nel sapere, nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

è l'acquisizione più rilevante. «Imparare ad imparare»: questa è la missione che la scuola deve rendere chiara agli studenti oggi. Di questo gli studenti avranno bisogno nella vita e questo la scuola dovrà offrire loro. Il nostro obiettivo, dunque, è costruire una scuola che non lasci indietro nessuno e che favorisca la mobilità sociale. Lo ha espresso molto bene la senatrice Carloni nel suo intervento. Occorre costruire una scuola che consenta di coltivare talenti, quale che sia la famiglia o il ceto sociale di provenienza. È un fatto di giustizia sociale, certo, di attuazione del principio costituzionale di uguaglianza, ma è anche un investimento necessario per la costruzione della società della conoscenza. Questa, signor Presidente, è la nostra filiera di valori: principio di uguaglianza, mobilità sociale, merito, società della conoscenza. In questo senso vanno il sostegno con le borse di studio a chi intende proseguire gli studi, l'elevamento dell'obbligo scolastico di due anni previsto dalla legge finanziaria fino all'investimento sugli asili nido. È noto, infatti, che le discriminazioni sociali sono l'effetto di scarsi investimenti in educazione nella primissima infanzia. A tal proposito, ricordo che abbiamo depositato un disegno di legge di iniziativa popolare, il quale prevede che l'asilo nido venga trasformato da servizio sociale a domanda individuale in servizio educativo

in linea con il principio educativo della continuità. Le sezioni primavera assicureranno una continuità fra il nido e la scuola dell'infanzia, rappresentando un passo avanti rispetto alla generalizzazione della scuola dell'infanzia e alla costruzione di una continuità da zero a sei anni.

per l'atteggiamento costruttivo sia della maggioranza che dell'opposizione, che ha consentito di migliorare il testo presentato dal Governo. Questa è la funzione del Parlamento.

E ha un valore enorme il fatto che la maggior parte degli emendamenti sia stata approvata all'unanimità. Al di là delle polemiche, colleghi dell'opposizione, questo è il fatto di maggiore portata, che qui dobbiamo valorizzare. Dunque, ringrazio ancora la relatrice, il Governo e tutta la Commissione per il lavoro svolto, per il bene degli studenti, dei nostri giovani e del sistema scolastico nel

Al di là delle posizioni politiche complessive in questa sede richiamate, il dibattito ha affrontato alcuni nodi cruciali con un'attenzione rivolta ad obiettivi comuni, talvolta con soluzioni diverse, peraltro anche all'interno della stessa opposizione e con qualche differente sensibilità perfino nella stessa maggioranza. Un dibattito vero. In ogni caso, abbiamo registrato una passione politica vera per la scuola, che corrisponde alla grande rilevanza sociale del tema di cui discutiamo, che è certamente un punto del sistema: non lo tocca tutto, ma è un punto significativo. È significativo in sé, per quello che viene prima dell'esame e per quello che accade dopo. Poi avremo modo, senatore Amato, di considerare, tutto intero, il contesto determinato dalla prossima legge finanziaria in materia di istruzione. Il primo punto emerso con chiarezza è quello della serietà, del valore dell'esame e degli studi, dunque della scuola. La collega Pellegatta ha richiamato il senso dell'equità. Se la scuola è seria, è più giusta. Questo significa rispetto per i ragazzi e per la scuola. E il senatore Valditara ci ha dato uno spunto di riflessione: qui è la contemporaneità, è la modernità. È moderno crescere responsabilmente. Diceva il senatore Asciutti che nell'immaginario pubblico c'è questa idea del tutti ammessi, tutti bravi, tutti promossi. Appunto, non va bene così.

Allora è più serio arrivare agli obiettivi indicati da questo disegno di legge. È serio togliere ossigeno ai «diplomifici». È più seria una commissione mista.

a destra, a sinistra e al centro di Benedetto Croce. Quanto al senatore Giovanni Gentile, richiamato questa mattina dal collega Strano, certo ha avuto un grande pensiero sulla scuola; ha avuto un grande pensiero della scuola collegata con la struttura della società, non solo sociale, ma anche politica. Eppure questo grande pensiero non ha impedito al Parlamento negli anni successivi alla sua riforma (1924, 1925 e 1926) di negare le libertà democratiche fondamentali. Noi capiamo cosa sia in gioco, non solo nel particolare, quand'anche decisivo e importantissimo, della scuola. Sono sempre in gioco la libertà e la democrazia del Paese. Il secondo,

abbiamo discusso anche sul senso dell'autonomia, sulla necessità che l'autonomia produca risultati e che questi siano comparabili sul piano nazionale e internazionale.

se tutti si debbono rimettere in gioco, che si rimetta in gioco anche l'Istituto nazionale di valutazione. Si tratta di arrivare alla misurazione concreta delle conquiste reali

delle responsabilità nazionali e dei livelli internazionali in cui vivono i nostri ragazzi. Il richiamo in causa di un invalsi rinnovato significa non pigrizia, significa non autoreferenzialità,

Ricordo che le ultime direttive del 2006, la n. 481 e la n. 2008, della Commissione europea sostengono la cultura della valutazione nei sistemi di istruzione come strumento necessario per promuovere i processi di modernizzazione dei sistemi di istruzione. Faccio notare come queste direttive prevedano anche finanziamenti per il raggiungimento di questi obiettivi. In terzo luogo, è emersa la discussione sul tema della parità scolastica; peraltro le obiezioni pregiudiziali di costituzionalità, già respinte da quest'Aula, hanno sollecitato un dibattito vero anche su questo È emerso con chiarezza che il provvedimento in esame si colloca su una strategia di fondo che ha due pilastri: la Costituzione e la legge n. 62 del 2000. C'è una grande storia nel rapporto tra sistema di istruzione statale e sistema non statale in questa conquista politica e democratica della parità scolastica. C'è il grande rapporto tra l'autonomia dei processi formativi, che sono sempre legati ad una forte esigenza della società civile, e, nello stesso tempo, la necessità di regole condivise, perché abbiamo bisogno di un sistema pubblico pubblico di istruzione che regga le sfide. Oggi il nostro sistema pubblico è costituito, come si sa, in gran parte di scuole statali, ma anche di scuole non statali. Sul tema, che ha visto l'attenzione di molti colleghi, vorrei dire semplicemente: in questo provvedimento gli esami di Stato incardinati nelle scuole paritarie sono posti nelle medesime condizioni di quelli delle scuole statali. Altro discorso - è qui la distinzione che vorrei fare - riguarda il tema dei commissari. I commissari esterni statali rispondono allo Stato e non vi è bisogno, a mio parere, di aggiungere altro. Questo è il senso vero di una serietà e questo è il senso anche di un ordine del giorno, che ho presentato e che è stato richiamato nella discussione, riguardante la formazione degli insegnanti e dei dirigenti che vanno a realizzare gli esami di Stato, formazione aperta al personale delle scuole non statali. «Aperta» vuol dire nel rispetto delle loro scelte e della loro autonomia, ma nella possibilità che si possa crescere insieme, con una stessa mentalità, che può

e per la sua equità, è un efficace sistema di istruzione pubblica, in cui forte sia la scuola statale e forte, nella sua iniziativa e nella sua autonomia, sia la scuola paritaria. Quello che importa, infatti, sono i risultati, i risultati di qualità; posto che abbiamo già riconosciuto, sulla scia della Costituzione, il senso della libertà e il senso della responsabilità, quando si istituiscono scuole statali e non statali. Ai colleghi Davico e Marconi vorrei dire che è necessario e urgente, se il profilo dell'esame di Stato è questo, mettere in moto le cose a conclusione di questo anno scolastico. Gli studenti l'hanno già capito e si sono già messi a studiare di più. *(Brusìo)*. PRESIDENTE Colleghi,

Quando, come dice la presidente Franco, è in gioco il futuro (e il futuro è già cominciato per i ragazzi), noi non possiamo accumulare altri ritardi. C'è infine l'idea di un raccordo molto forte, di sistema, tra l'istruzione secondaria superiore, gli esami di Stato, l'università, la formazione superiore, perché appunto si acquisisce qui quello che ormai, nelle dichiarazioni ufficiali

richiamando l'idea che i ragazzi, per quello per stiamo discutendo e per la nostra responsabilità, sono anche un bene pubblico; lo sono in ogni parte del Paese, al Sud come al Nord. La scuola deve avere la capacità di dimostrare che il suo significato è

al Ministro e alla vice ministro Bastico, perché raccolgano tutti gli stimoli del dibattito e ne tengano conto anche nelle loro direttive future per l'attuazione della legge. Insomma, è stato qui evocato un nuovo spirito della scuola italiana; è come

capirli, rispettare le loro emozioni, rovesciare la logica, fare dell'esame non una costrizione ed uno spauracchio, ma un'opportunità, in modo che la paura si trasformi anche in soddisfazione. Anche così, infatti, i nostri ragazzi saranno messi nelle condizioni di capire meglio la vita. Non posso concludere questa replica, signor Presidente, senza andare col pensiero a ciò che è accaduto in questi giorni come un fatto emblematico; profonde inquietudini attraversano il percorso scolastico dei nostri ragazzi e non possiamo pensare che una legge e un esame di Stato siano quei meccanismi universali che mettono a posto le cose. Mi riferisco alla vicenda

che in queste condizioni non hanno affatto superato l'esame della vita, che la prima pietra della cultura è l'umanità e il rispetto dell'altro e che finché accadono cose come queste un altro esame attende la scuola e tutti noi? Ma che Paese ormai sta diventando l'Italia se tollera un *humus* di questo genere! Allora, oggi dobbiamo ricavare questo segnale nel vivo della vita del Paese: cultura ed educazione, educazione e cultura; una scossa morale, insomma, insieme con le leggi

e di cui sono grata davvero a tutti.

anche agli onorevoli senatori per l'ampio, argomentato e alto dibattito che hanno proposto in quest'Aula e per il lavoro approfondito, puntuale e serio che è stato svolto in Commissione. Ringrazio in particolare la senatrice Soliani, relatrice del provvedimento, e la senatrice Vittoria Franco, presidente della 7a Commissione permanente, che sono stati due riferimenti fondamentali per lo svolgimento di questo importante lavoro. Questo impegno testimonia l'attribuzione di un'importanza fondamentale, oserei dire, di un punto di centralità al tema dell'esame di Stato. Una centralità che, in effetti, questo tema merita e che il Governo ha voluto sottolineare con la presentazione del primo progetto di legge in tema di istruzione, proprio sull'esame di Stato. L'esame di Stato è quello che rilascia il titolo di studio finale di un percorso di studio e costituisce quindi il riconoscimento per il ragazzo del percorso di studio che ha effettuato e della sua serietà e costituisce anche, per lui, il titolo di accesso ad un percorso lavorativo, professionale

è stato segnalato come nessuna autorevole università nel nostro Paese consideri più l'esito dell'esame di Stato come elemento di accesso agli studi e di valutazione.

lavoro. Facciamo una scelta per superare questa deriva che porta progressivamente al superamento del valore legale del titolo di studio. Noi non vogliamo questo superamento, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista dei fatti. Vogliamo che l'esame rilasci un titolo di studio significativo a compimento di una scuola che vogliamo progressivamente modificare nell'ottica così efficacemente illustrata dalla senatrice Carloni: una scuola inclusiva,

Da questi obiettivi traggono la loro origine una serie di norme contenute nel progetto di legge, strumenti coerenti per dare più credibilità ed autorevolezza all'esame di Stato. del ripristino della commissione mista con il Presidente esterno; del ripristino dello scrutinio finale con un giudizio di ammissione; del recupero dei debiti contratti negli ultimi tre anni (norma, questa, che entrerà progressivamente in vigore);

La senatrice Negri ricordava il numero elevatissimo di privatisti e soprattutto la progressione velocissima, verificatasi in questi ultimi anni, del loro numero. Vogliamo dire con grande chiarezza ai ragazzi che in queste norme non c'è alcun criterio punitivo. Al contrario, c'è la valorizzazione di sacrifici e impegni attuati nel *cursus* scolastico. Vogliamo anche evidenziare che è a loro garanzia e tutela che queste norme sono proposte all'approvazione del Parlamento.

Noi intendiamo operare un processo complessivo di cambiamento. Quindi, anche questo progetto di legge di modifica, che costituisce un passo avanti di grande importanza e significato, a nostro avviso sugli esami di maturità,

Nella finanziaria è prevista una norma di modifica radicale della *governance* complessiva dell'INVALSI, cui sono già state inviate direttive puntuali per una modifica totale dell'attuale sistema di valutazione.

in avanti importante. L'INVALSI fornirà schede e modelli di riferimento che le autonomie scolastiche potranno scegliere. Confermo che l'autonomia deve costituire un valore fondamentale di riferimento nella

come strumenti per la valutazione degli apprendimenti e dei saperi dei ragazzi, coerentemente con le modalità valutative di carattere internazionale ed europeo, costituisce un importante passo in avanti ed una scelta della Commissione di grande significato.

che i candidati esterni non possono accedere alle scuole paritarie, perché così recita esattamente il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo Ecco, abbiamo applicato la legge n. 62 del 2000, ma vi abbiamo inserito delle norme correttive, perché andare in una scuola paritaria non può costituire la scorciatoia per il privatista per avere un esame facilitato: da qui

per affrontare un tema per noi importantissimo: aumentare la collaborazione tra scuola e università. Ci sono norme importanti sull'orientamento da svolgersi già nella scuola per i percorsi di studi successivi al termine degli studi superiori. Ci sono, ancora, elementi importanti per la valorizzazione dei percorsi di istruzione e dell'esito finale dell'esame di Stato. Ricordo che abbiamo introdotto in un emendamento anche l'elemento della lode per valorizzare ulteriormente le abilità. Vi sono ovviamente norme che rafforzano l'intreccio, la collaborazione tra le due autonomie, quella scolastica e quella universitaria, nel rispetto pieno del valore costituzionale dell'autonomia scolastica e dell'autonomia universitaria.

emendamenti che, anche ad avviso del Governo, costituiscono un miglioramento rispetto al testo iniziale. Lo abbiamo reso coerente, con la convinzione che il miglioramento della scuola, dell'università, dei sistemi della formazione costituisce una priorità fondamentale che deve coinvolgere tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, le forze sociali e professionali del nostro Paese. Il Governo, per quanto sarà di sua competenza, farà di tutto perché il confronto sia reale, di merito e costruttivo: solo così possiamo far fare alla scuola quei passi in avanti, di miglioramento e di riforma, riforma, indispensabili per il nostro futuro. «Scuola, scuola, scuola» hanno richiamato in questi giorni molti autorevoli commentatori, sia partendo dai drammatici e tragici eventi accaduti in questi giorni, già ricordati dalla senatrice Soliani, sia richiamando le prospettive del nostro Paese. voglio qui richiamare l'autorevole intervento del Governatore della Banca d'Italia. E allora se «scuola, scuola, scuola» è, siamo impegnati tutti affinché questo avvenga con la massima collaborazione e con la massima condivisione delle scelte.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, preso atto del recepimento delle condizioni poste alla Commissione di merito ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.25, 1.26, 1.46, 1.165, 1.169, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185 e 1.317, nonché parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.510 e 1.35. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti esaminati».

il disegno di legge n. 960 persegue l'obiettivo di modificare le norme che regolano gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, contenute nella legge 10 dicembre 1997, n. 425. All'articolo 4 il disegno di legge governativo prevede infatti il ripristino della composizione mista delle commissioni d'esame, con non più di sei commissari, di cui il cinquanta per cento interni e il restante più un presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni o classi. I soggetti destinatari della nomina a commissario esterno all'istituto e a presidente sono scelti tra coloro che provengono «esclusivamente» dagli istituti di istruzione secondaria superiore statali.

ritenendo, peraltro, che le predette potessero sfociare, nell'altro ramo del Parlamento, in una questione pregiudiziale di costituzionalità. Ribadisco con vigore che le scuole paritarie fanno parte quanto quelle statali del sistema nazionale, tant'è che esse sono abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale. Per quanto attiene ai docenti, ribadisco ulteriormente che l'attuale sistema di reclutamento dei docenti prevede il doppio canale, vale a dire quello dei cosiddetti concorsuati e quello dei cosiddetti precari storici. Le assunzioni avvengano per il 50 per cento attingendo alle graduatorie di merito, costituite da docenti che hanno partecipato al concorso ordinario, e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti, delle quali fanno parte sia i docenti che hanno superato il concorso ordinario, sia quelli che hanno partecipato ai corsi abilitanti riservati, ed infine i cosiddetti SSIS. Fatta eccezione per quella piccola quota di docenti che prestano servizio sotto forma di volontariato o con contratti di prestazione d'opera, posseggono anch'essi una posizione giuridica identica a quella detenuta dai docenti delle scuole «statali». In caso contrario, i docenti delle scuole paritarie non potrebbero far parte delle commissioni degli esami di Stato, in veste di commissari interni (come già avviene, da sempre). Restando forti le riserve di carattere incostituzionale dell'articolo 4 del disegno di legge n. 960, anche alla luce delle normative vigenti in materia di formazione di graduatorie e assunzione di personale docente nelle scuole, avanzo la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 960, così come previsto dall'articolo 96 del Regolamento del Senato. Presidente, che il voto sulla proposta che ho appena illustrato sia anticipato dalla verifica del numero legale in Aula.

all'esame degli articoli, non solo perché l'ampio dibattito, le controdeduzioni della relatrice e infine l'intervento del vice ministro Bastico

per la crescita del nostro Paese. Ci sembra davvero poca cosa l'argomentazione addotta, per cui un Governo qualifica la propria azione nel settore della scuola proprio partendo dagli esami, perché da essi si possa qualificare tutto il percorso. Ci sembra davvero poco che il Governo si presenti in Aula con il primo provvedimento che riguarda la scuola e non avverta minimamente la necessità di rendere noto a quest'Aula quale sia il percorso complessivo che intende che intende seguire nella realizzazione di una politica per la scuola. Debbo davvero rilevare come la precarietà politica di questo Governo stia animando anche un dibattito che dovrebbe essere fondamentale. Forse la rappresentante del Governo avverte questa precarietà, forse la rappresentante del Governo non si sente di dare indicazioni di prospettiva, di dare a quest'Aula indicazioni di percorso, proprio perché della precarietà questo Governo ha fatto il filo conduttore in tutte le branche dell'amministrazione che dovrebbe portare avanti. E allora in questo scenario, in un momento così delicato proprio dal punto di vista della programmazione finanziaria della vita dello Stato, si viene qui a dirci che la priorità è costituita dal fatto che dobbiamo riformare gli esami di Stato. Non parliamo dei fenomeni di bullismo emersi proprio questi giorni, non parliamo delle esigenze di dotazioni finanziarie, non parliamo della motivazione che debbono avere gli operatori della scuola. Suonano come offensive le parole contenute nella relazione al presente disegno di legge, in cui si dice che bisogna modificare gli esami di Stato perché la classe docente ha ritenuto in questi anni di essere quasi autoreferenziale. Una classe docente di cui si parla in termini negativi e non in termini propositivi: non si parla di incentivare l'entusiasmo della classe docente, non si parla di collaborazione, di sinergie che devono essere trovate nel mondo della scuola, ma soltanto di ciò che dev'essere la selezione finale dello studente. Non si parla dello studente come futuro cittadino, non si parla dello studente come competitore in Europa rispetto alla creazione di nuovi modelli di sviluppo, non si parla di protagonismo del giovane d'oggi rispetto alle sfide del futuro: si parla di un esame che deve essere più selettivo, ma per giungere a tale selezione

ci sembra troppo poco e davvero deludente che si possa affrontare un argomento così delicato partendo dalla fine, senza ricondurre tutto il percorso alla coerenza. Il passaggio alla disamina dei singoli articoli un fatto che riteniamo davvero superfluo, in un fase in cui ancora non abbiamo visto disegnare una politica per la scuola. Ci sembra davvero superfluo e una perdita assoluta di tempo, perché sappiamo che questo provvedimento non aggiungerà nulla alle potenzialità che devono avere i nostri giovani. Il provvedimento in esame non darà nulla

Come fa, senatrice Soliani? Anche lei, come autorevoli rappresentanti di questo Governo, partecipa a sedute spiritiche che riescono ad informare anche sulle intenzioni dei nostri studenti?

diversa e stigmatizzo anche il comportamento: Parecchie scuole italiane e parecchi giovani hanno tratto occasione da questo provvedimento per marinare qualche giornata di scuola.

senatore Amato).* Noi, classe dirigente di questo Paese, possiamo ridurre e ricondurre la politica scolastica soltanto a una vendetta postelettorale? Intendo bene che questa maggioranza ha cambiali da rendere all'incasso. Questa maggioranza ha più che altro la smania, anche perché ormai è l'unico collante politico che la sostiene, di poter dire che ciò che di vagamente berlusconiano c'è stato in qualunque riforma del nostro Paese deve essere demonizzato prima e demolito subito dopo. Ma avete iniziato dal lato sbagliato e col piglio sbagliato. Avete voluto dare dalla coda l'idea di quello che sarà il corpo del mostro che creerete nel settore della scuola. In un precedente intervento di un collega della maggioranza è stato sostenuto che questa è una casa che si costruisce stanza per stanza. Ma se l'architetto o il costruttore non ha ben chiaro in mente come deve essere la casa da costruire, casa ad avere alla fine un assetto armonico e, soprattutto, utile alle esigenze delle nostre nuove generazioni? Come potete costruire stanza per stanza, senza sapere qual è la casa che volete dare agli studenti del nostro Paese?

che direzione volete far prendere in tutti i settori: economico, sociale e anche di politica comunitaria. Ma sui ragazzi no, questo *non* *licet*: non è lecito che sul futuro dei giovani possiate andare a tentoni e continuare, con scelte demagogiche e populistiche di natura elettoralistica, a scherzare senza

avendo in mente tutto il progetto. In questa casa metteremo il nostro mattone, ma con responsabilità e avendo fiducia nel futuro del nostro Paese e nei nostri giovani.

1.47 chiede di sostituire al comma 1, la lettera a), in maniera tale che i debiti formativi contratti dai singoli studenti siano sì saldati, ma dietro una regolamentazione nazionale per evitare che ogni singola istituzione possa stabilire le proprie modalità.

in modo che i nostri studenti possano essere ammessi solo se abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle lezioni. Nel testo dalla Commissione, in realtà, la presenza, la partecipazione alle lezioni non è minimamente prevista. Almeno, si parla da parte della relatrice, da parte del Governo di rigore sull'esame conclusivo, ma non si attua un minimo di rigore nella partecipazione degli studenti alle lezioni.

1.165 si illustra da solo.

a domande, risposte. Non ci interessa se l'alunno ha le competenze che oggi la società moderna e l'Europa ci chiedono.

ma un credito scolastico eccessivamente pesato, si presenti agli orali senza avere bisogno di alcun voto, perché ha già raggiunto il minimo per il superamento dell'esame. Non faremo il bene dello studente, dando un peso eccessivo al credito scolastico. 1.164, ribadisco il problema delle commissioni. Signor Presidente, nel 2001

che hanno adottato il loro piano dell'offerta formativa sanno su cosa valutare, conoscono i loro studenti e non incorriamo nel meccanismo perverso della «vendita» delle lezioni private tra una scuola e l'altra.

Noi parliamo di insegnanti collocati a riposo:

fare i membri esterni, essendo anch'essi parte del servizio pubblico nazionale, sia perché si evita, inoltre, che un supplente temporaneo non abilitato possa partecipare come commissario esterno agli esami di Stato:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato pochi emendamenti, abbiamo presentato pochi emendamenti, ma tutti qualificati, tutti su punti fondamentali, di sostanza e non dunque emendamenti di semplice contorno.

I nostri emendamenti sono tutti espressione di valori di riferimento: il valore della serietà, quello della responsabilità, quello del merito, quello della libertà educativa, quello dell'autonomia.

e Ranieri, ma anche a senatori che in passato si sono sempre dichiarati favorevoli ad una valutazione del sistema scolastico, come il senatore Fisichella.

che ha votato solo per spirito di obbedienza e di rispetto ad una disciplina più generale di maggioranza - questa sia una grande occasione per capire chi veramente vuole un rinnovamento e una modernizzazione della nostra scuola, una scuola autonoma, ma anche responsabile, e chi vuole iniziare a concepire una valutazione delle nostre scuole non soltanto come verifica della preparazione dei nostri studenti. Credo che l'emendamento 1.21 sia un po' la cartina di tornasole per comprendere la bontà di ciò che si dice.

far crescere la nostra scuola e per ripensare complessivamente il nostro modello di scuola all'insegna di quel valore di serietà che è stato così tante volte richiamato negli interventi, ma che poi deve trovare testimonianza concreta nelle singole votazioni.

pur non essendo favorevole alla revisione dell'attuale normativa sugli esami di maturità, abbia preso in seria considerazione i disegni di legge presentati dal Governo e dai senatori Valditara, Schifani e Asciutti, cercando di dare un contributo propositivo e costruttivo. Non abbiamo scelto né una linea rigorista né una linea del tutto permissivista, tutta a favore del pubblico o tutta schierata ciecamente a favore delle scuole private. Abbiamo cercato, con sano buon senso, liberi da qualsivoglia visione ideologica, di cercare soluzioni concrete ai mali che, di volta in volta, si sono manifestati nell'applicazione di questa tormentata normativa che, come ricordato in più di un intervento, è stata fin troppe volte modificata negli ultimi quindici anni. E proprio perché le visioni politiche si sono contrapposte e fronteggiate, desideriamo che questa non sia più una materia di scontro, terreno nel quale ritrovare e cercare la rivincita sull'avversario. Desideriamo piuttosto, con uno sforzo di equità

È vero che l'esame di maturità è diventato negli ultimi anni qualcosa di poco significativo, di troppo leggero, e che non ci si prepara più in vista di esso con la dovuta serietà. In una parola, potremmo dire che l'esame non tira più come una volta quella volata di intensità di studio, di approfondimento e di slancio che fa parte di una maturazione seria nella vita di una persona. Se concepito in questa logica, e non in quella dell'esame che serve a bocciare, possiamo anche condividere la necessità di introdurre elementi che si spera possano servire, non ad aumentare l'angoscia dell'esame, ma un serio e sereno stimolo per presentarsi di fronte ad un appuntamento con la ferma volontà di superare la prova. In questo senso i nostri emendamenti. Certamente quello che vuole allargare a tutti gli anni di corso il contenuto del colloquio. Non deve essere un esame particolareggiato, ma credo che non sia scandaloso verificare se un giovane del liceo classico abbia un'idea approssimata dei secoli nei quali Roma è stata monarchica, repubblicana o imperiale. Come credo non sia punitivo scoprire in un candidato di liceo scientifico le basi della matematica e della geometria attraverso un ragionamento elementare. Ma al tempo stesso non vediamo per nulla male, anzi la l'opportunità per chi abbia conseguito una qualche insufficienza di poter essere ammesso all'esame. Infatti questa modalità è consentita in tutti gli anni precedenti. Creare a valle uno sbarramento che impedisca di passare in questo modo è profondamente ingiusto. Non andrebbe consentito neanche prima. Dovrebbero essere ripristinati gli esami di riparazione a settembre, una logica che non mi sembra sia più condivisa da nessuno. nessuno. Con questa nostra proposta l'esame acquista un reale significato aggiuntivo: per i più deboli, quelli che hanno trascinato malamente la loro carriera scolastica per tutto il quinquennio, la possibilità dell'estremo appello per potere concludere il ciclo degli studi; per chi ha invece superato brillantemente ogni anno di corso la doppia opportunità, o di scontarsi un anno intero o di accedere agevolmente all'esame con una quota significativa di crediti, che vogliamo aumentare rispetto al colloquio, che vanno ad incidere sul voto finale e la possibilità di quelle «eccellenze» che ammetterebbero lo studente con particolari meriti, riconosciuti formalmente nel mondo del lavoro o dell'università. In verità, sempre nella direzione di premiare il percorso didattico complessivo, abbiamo anche proposto, con il collega Buttiglione, di diminuire il punteggio per i colloqui e di aumentare quello per la valutazione dei crediti. Al riguardo vorrei aprire una breve parentesi su quello che ritengo un singolare ordine del giorno votato in Commissione e già accolto dal Governo, tanto che non viene ripresentato in Aula. Ebbene, in questo si impegna il Governo, appunto, ad «impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro». In mezzo a tanto rigore e volontà di dare all'esame un valore di svolta profonda, che di per sé non potrà mai avere, si inserisce questa amena disposizione che consente al giovane candidato di fare una chiacchieratina sul suo futuro,

E' questo aspetto che appare singolare e lievemente preoccupante. Una prassi di questo tipo era già in uso quando sostenni, ormai qualche decennio fa, l'esame di maturità,

Farlo diventare norma, introducendo una facoltà riconosciuta, mi sembra eccessivo e rischia di diventare una distrazione anche ai fini della stessa valutazione. A cosa serva questa disposizione, a quale *ratio* risponda, non sono riuscito a capirlo. Mi sembra che risponda alla logica del "tutto e un po' di più" contenuta in questa riforma, frutto e risultato di successive sovrapposizioni e stratificazioni legislative. Comunque, resto contrario all'idea che un candidato parli in modo formale dei suoi progetti futuri. Il farlo condizionerà inevitabilmente chi ascolta in senso positivo o negativo; e far entrare le scelte libere e personali di un giovane nell'esame di maturità mi sembra un po' eccessivo. Non vorrei lanciarmi in facili ed ironici esempi, ma come giudicherebbe una commissione di pacifisti un giovane candidato che vuole partire volontario per l'Afghanistan o per altra zona di intervento militare deciso dal nostro Paese? Quale accoglienza riceverebbe una giovane che dichiarasse di scegliere la clausura religiosa appena diplomata, di fronte ad una commissione composta da ferventi atei laicisti? Questa disposizione rischia di innescare inutili ed ipocrite sceneggiate o - spero in casi rari - antipatiche discriminazioni. Comunque, la eviterei e spero che il Governo non ne faccia alcun uso significativo. Altri emendamenti riguardano la possibilità per i docenti delle paritarie di partecipare alle commissioni come esterni e la non applicabilità della legge nel corso dell'attuale anno scolastico. Un ultimo accenno a favore della proposta di estendere all'intero territorio nazionale il reclutamento dei commissari di esame, preferendo quelli più vicini alla sede, dell'altra che tende a stabilire che l'INVALSI non fornisca appena i modelli per la terza prova, ma fornisca i testi contenenti gli argomenti da porre a disposizione delle autonomie scolastiche.

Presidente, l'illustrazione degli emendamenti da noi presentati si può racchiudere in tre argomenti, in tre capitoli, più una visione generale che abbiamo sull'intero sistema scolastico. Noi pensiamo - ed abbiamo invitato in questo senso il Ministro, la prima volta che è venuto in Commissione a relazionarci sulle linee programmatiche del suo Ministero - che il Ministro non debba essere solo Ministro della scuola o dell'istruzione pubblica, come una parte della parte che governa il Paese in questo momento vuole che sia; noi pensiamo che la scuola vada pensata pensata in termini moderni, che non sottintendono comunque il valore sociale, culturale e politico che la scuola deve avere. Tale valore consiste nel far crescere tutta la popolazione, partendo - è questo il servizio di Stato fondamentale, fondamentale, storico, che va riconosciuto - da chi è in situazione di maggior debolezza, ma senza impedire che chi non è in queste condizioni di maggior debolezza e che quindi può, in qualche modo, accedere a livelli di istruzione o a percorsi differenziati per capacità, per cultura, per intelligenza o per tanti altri motivi, senza impedire, insomma, a chi può fare di più di fare di più. Quindi, bene l'idea di partire e di creare un sistema che aiuti tutti, che dia il necessario e l'essenziale per tutti, anche in senso nazionale, se vogliamo; ma non si può impedire a chi può fare di più, anche per appartenenza territoriale, di fare di più. A volte alla scuola si chiede e si deve chiedere anche di più. Avevo pertanto invitato il Ministro, in quell'occasione, ad essere non il Ministro della scuola di Stato,

del 68. L'articolo 68 della finanziaria è quello che interessa la pubblica istruzione. Il Ministro ci ha riportati al '68 se vogliamo; può essere una battuta, ma può anche essere intesa in senso culturale e politico. Quindi, in questo senso non bisogna avere paura della modernità perché bisogna coniugarla con quella che è la tradizione più forte e importante del nostro Paese relativa alla scuola.

un coordinamento, di fare sistema di tutto l'apparato della formazione e dell'istruzione. Quindi c'è la scuola di Stato, c'è la scuola non di Stato, paritaria, c'è anche la scuola privata; mica bisogna spaventarsi di questo. Ci sono anche studenti che vanno a scuola all'estero,

State fermando anche in questo senso il Paese, state fermando anche in questo senso il progresso, state fermando e impedendo al nostro sistema scolastico di essere europeo; quell'Europa che tutti sbandierano, che tutti manifestano, con cui tutti si sciacquano la bocca, ma che alle è un'Europa lontana, che ha già fatto e sta facendo molti passi in avanti rispetto a noi. Ciò soprattutto e a partire dal sistema scolastico e da quello formativo che - ripeto - deve essere realizzato dal sistema dello Stato, dalla scuola dello Stato, dalla formazione professionale delle Regioni, da tutte le componenti che ci possono essere. In questo senso molti dei nostri emendamenti e dei nostri articoli si riferiscono alla possibilità

L'altro grande tema è quello della serietà; in questa riforma, in questo nuovo esame c'è qualche barlume e qualche tentativo di serietà. Tuttavia, essi non bastano ancora perché resta aperto il sistema della della chiusura e della soluzione dei crediti formativi dei ragazzi. Abbiamo infatti - non nascondiamocelo - ragazzi che effettuano tutto il percorso scolastico senza sanare i loro debiti e quindi arrivano all'esame con qualche punticino in meno, ma in meno, ma l'impostazione che è stata data non risolve il problema. Chiunque può arrivare all'esame pur non avendo saldato i debiti degli anni precedenti. Non possiamo ridurre l'esame a schede con quiz, con domande chiuse, con semplificazioni delle materie legate

tutto decade, quella serietà che si cerca alla fine non la si trova. Quindi abbiamo stabilito un numero che è di sessanta giorni sui circa duecento di scuola. Perché i ragazzi, sempre per il discorso di serietà che facevo prima, siano valutati correttamente e coerentemente pensiamo che i migliori commissari debbano essere i membri interni, coloro che li hanno seguiti, portati avanti, fatti crescere, che

maggiore serietà cercata, queste norme che vanno ad irrigidire il sistema, queste nuove richieste di di maggiore impegno, di superamento di prove preliminari, di saldo dei debiti non possono e

alla possibilità di inserire una terza prova a carattere pluridisciplinare, predisposta a norma di legge dall'INVALSI.

sulle quali verterà l'esame. Secondo noi, però, è altrettanto importante che i professori posseggano completamente le qualità per insegnare ai nostri ragazzi. Siccome è necessario stabilire se, alla fine del ciclo di studi, lo studente abbia raggiunto un risultato appagante per se stesso e per la società che dovrà

Tali emendamenti mirano ad affermare che i privatisti e i candidati esterni devono presentarsi a sostenere gli esami solamente nelle scuole statali. Questa posizione non è dettata da una logica statalista e centralista. In realtà, vogliamo cogliere gli elementi di novità e di riflessione sul rapporto pubblico-privato che le culture democratiche, attente alla trasformazione delle istituzioni, hanno oggi posto in campo su questa relazione. Rifondazione Comunista ha portato avanti una battaglia parlamentare, in opposizione alla legge n. 62 del 2000, la cosiddetta legge di parità, che avrebbe dovuto, secondo il dettato costituzionale, assicurare agli alunni delle scuole non statali un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (quarto comma dell'articolo 3 della Costituzione). A questa legge che sul finanziamento pubblico ha comunque aggirato i vincoli costituzionali e contro la quale abbiamo, anche insieme ad altre forze, politiche e sociali, promosso due *referendum* regionali, oggi ci riferiamo con spirito repubblicano, pretendendo dal Parlamento la fedeltà al suo testo. All'articolo 2, questa legge definisce i caratteri di tale parità, quando in stabilisce che le scuole paritarie hanno l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Ebbene, questo è il punto: i candidati esterni non sono paragonabili ed equiparabili agli alunni delle scuole paritarie, proprio perché non ne sono alunni, cioè non le hanno frequentate. Ci troviamo di fronte, insomma, a una forzatura, a un'interpretazione estensiva di questa legge di parità, in un tentativo tutto ideologico e politicista che porta a una duplice incongruenza giuridica. le scuole paritarie private in questo modo rilascerebbero certificazioni aventi carattere legale al di fuori della platea loro naturale, cioè al di fuori degli alunni loro iscritti. Solo in rapporto a questa platea esse possono esercitare tale funzione che la legge di parità attribuisce. Seconda incongruenza giuridica: si confonde l'esercizio di una funzione pubblica esercitata nelle scuole paritarie verso i propri iscritti con il carattere, o meglio, la natura di queste scuole, che è appunto privata. Una funzione può essere attribuita ma non si può trasmettere il carattere e la natura pubblica a ciò che si definisce privato per scelta costitutiva. Le scuole paritarie private non sono istituzioni statali o articolazioni dello Stato, quindi quando esercitano la funzione di rilasciare diplomi la possono esercitare non *erga* *omnes*, ma solamente rispetto ai propri alunni.

Tale sensibilità va giustamente rappresentata e messa a valore nel dibattito pubblico, quindi in Parlamento. Del resto, questa posizione, che è laica e tenacemente legata alle ragioni costitutive della scuola pubblica, per nessun motivo può essere segno di divisione interna alla coalizione o di interesse di parte oppure di debolezza della nostra alleanza politica.

in modo surrettizio una modifica di portata, a mio parere, istituzionale nel rapporto scuola pubblica-scuola paritaria. pertanto tutti le senatrici ed i senatori che hanno seguito il filo di questo ragionamento, proprio per amore della laicità e dell'applicazione delle leggi che questo Parlamento ha approvato,

Presidente, gli interventi già svolti dal senatore Valditara e dal senatore Delogu...

Dal caos raggiungiamo l'ordine nuovo, l'essenza del futurismo che fa parte della nostra radice. Lei si rivolge al papalismo, noi ci rivolgiamo al futurismo; sono due concezioni diverse della vita. *(Applausi dal

Il mio intervento è teso soltanto a rilevare come i nostri emendamenti si rifacciano ad una concezione della scuola che ho già

brevemente per illustrare l'emendamento 1.315, l'emendamento 1.315, che salvaguarda le modalità di svolgimento dell'esame di maturità nella Regione autonoma della Valle d'Aosta quanto alla tipologia e alle modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova in lingua francese, in aggiunta alle tre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Questa situazione di fatto ha sancito definitivamente le modalità di svolgimento le modalità di svolgimento della quarta prova in lingua francese in attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare - la cui composizione sarà pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna è convocata, per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mercoledì 15 novembre 2006 alle ore 14,15 presso il Palazzo di San Macuto. **Interpellanze